Grazie

è certamente con piacere che torno oggi a informare il Senato sugli ultimi sviluppi della situazione nei Paesi del Mediterraneo, anche alla luce di una recente visita che ho compiuto in alcuni Paesi chiave nella sponda sud-mediterranea e dei contatti che ho tenuto nel corso delle due settimane che ci separano dall'ultimo incontro avvenuto qui, dinanzi a voi. Certamente sapete le dimensioni del fenomeno migratorio che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni e conoscete le caratteristiche del flusso e i dati che sono stati pubblicati dal Ministero dell'interno. È forse utile ricordare che nelle ultime ore, oltre al numero, ormai fortunatamente stabilizzato, da almeno 24 ore, di immigrati tunisini, le nostre forze di polizia hanno intercettato delle organizzazioni e dei gruppi di immigrati che stavano cercando di entrare clandestinamente nel territorio nazionale, in alcuni casi via terra: una cinquantina tra cittadini afgani e cittadini iracheni nascosti in alcuni TIR. Questo è quanto è avvenuto ieri. stato un tentativo a bordo di una barca a vela e sono stati arrestati due scafisti greci: nuovamente, clandestini afgani, iracheni e - in qualche caso - iraniani.

e iraniani che stavano cercando di approdare alle coste calabresi di Isola di Capo Rizzuto. Infine, un numero

una motovedetta della Guardia di finanza, ma è stato accertato con grande chiarezza che a bordo di quel barcone vi erano altri tre

a proseguire sulla strada di questa che potremmo chiamare una rivoluzione pacifica, ossia sul cammino delle riforme, della democrazia e verso le elezioni che si svolgeranno non oltre il prossimo mese di agosto. Il Primo Ministro tunisino mi ha parlato di iniziative importanti, anche di tipo legislativo: la Tunisia sta

Convenzioni internazionali sulla difesa e la protezione dei diritti umani, in particolare la Convenzione contro la tortura quella che ha istituito la Corte penale internazionale. Sono tutti segnali della volontà del Governo transitorio tunisino, che sosteniamo fortemente, di entrare in un quadro normativo internazionale che garantisca il pieno riconoscimento dei diritti. Abbiamo parlato a lungo anche delle caratteristiche del Governo transitorio tunisino che è composto in parte consistente da personalità di grande reputazione nella società civile, in alcuni casi

che da parte del Governo tunisino sono arrivate alcune importanti dichiarazioni di impegno politico: la prima è il forte impegno del Governo Ghannouchi a contrastare con ogni strumento legale il traffico degli esseri umani. Era questo un impegno che ci attendevamo fortemente e che ha trovato nella risposta del Primo Ministro tunisino un segnale soddisfacente, a mio avviso, della volontà effettiva di contrastare questo fenomeno drammatico. Sapete che nei giorni della grande ondata migratoria dalla Tunisia (oltre 5.000 persone in pochi giorni) si erano verificate situazioni di vera e propria lista d'attesa, con pagamento di somme rilevanti per ciascuna di queste che sono in realtà vittime di un traffico orribile, e che pagavano dai 1.000 ai 1.500 dollari a senza alcuna garanzia neanche di sopravvivere durante la traversata. È avvenuto in qualche caso il tragico naufragio, con la morte di immigrati che stavano arrivando verso le coste italiane. Il punto vero è la consapevolezza politica che noi abbiamo colto nel Governo tunisino che il traffico degli esseri umani è qualcosa che non solo danneggia in modo orribile persone, che sono assolutamente delle vittime, ma danneggia fortemente il sistema Paese della Tunisia, il sistema economico, perché in molti casi quel flusso di traffico di esseri umani, ben organizzato - bisogna dirlo - priva il Paese di potenzialità, di risorse umane importanti. Tra gli immigrati arrivati in Italia ovviamente ci sono anche persone, in una percentuale che non siamo in grado di verificare ancora, ben istruite, ben educate, con un livello professionale importante, che quindi è sottratto al loro Paese. Tunisi ha reagito, da subito, dopo la mia visita dell'altro ieri sera. Ha schierato le forze di sicurezza lungo la costa tunisina, proprio in prossimità dei porti da cui le partenze si erano verificate, i tre porti principali di Gabes, Sfax e di Zarzis,. Sono stati fermati ai porti di partenza almeno

di attuare una collaborazione molto forte con la Tunisia, una collaborazione italiana e soprattutto europea. Vi sono delle iniziative bilaterali, di cui ovviamente abbiamo parlato. Esiste un accordo italo-tunisino in vigore da anni, che non era stato pienamente attuato e che - lo abbiamo saputo dalle agenzie ieri - il Consiglio dei ministri della Tunisia ha ripreso in mano per valutarne l'immediata messa in applicazione, secondo delle regole e dei principi che noi avremmo auspicato. Ho espresso al primo ministro Mohamed la volontà del Governo italiano di mettere a disposizione uomini e mezzi della missione Frontex, che l'Europa si è già detta disponibile a far partire con immediatezza. Ed ho fatto appello alle forze tunisine affinché, per quanto riguarda le loro acque territoriali, possano collaborare con la missione internazionale Frontex, in modo da costituire un sistema di prevenzione alla partenza dai porti tunisini, aiutando così il pattugliamento in acque internazionali che, come sempre, è compito di Frontex e dell'Unione europea. Abbiamo chiesto di convocare con urgenza delle iniziative europee. La risposta è stata positiva. Domenica ci riuniremo come Ministri degli esteri per fare il punto non solamente sulla Tunisia, ma anche sulle politiche di partenariato e di vicinato dell'Europa con i Paesi del Mediterraneo. Il successivo mercoledì si riuniranno i Ministri dell'interno per le decisioni operative. Nella settimana vi sarà la decisione operativa della partenza della missione Frontex. Attendiamo che, anche su richiesta del Presidente del Consiglio europeo, si possa avere una sessione speciale dei Capi di Stato e di Governo dedicata al tema del Mediterraneo, affinché l'Europa ponga una visione strategica di medio e lungo termine, e non si limiti alla gestione dell'emergenza. L'Italia ha presentato un documento articolato: sono otto punti dettagliati di richiesta del nostro Paese alla Commissione europea. documento riguarda l'azione di prevenzione, la reazione e i pattugliamenti, il finanziamento per venire incontro, almeno in parte, alle spese aggiuntive che l'Italia dovrà sopportare per questo. Ma, con una visione più ampia, sto preparando un documento strategico che presenteremo domenica ai Ministri degli esteri, che

per la sicurezza e per la prosperità. Abbiamo registrato il sostanziale fallimento dell'Unione per il Mediterraneo - bisogna ammetterlo - ma è evidente che l'Europa non si può sottrarre al suo dovere di rilanciare la politica mediterranea, e l'Italia non si può e non si deve sottrarre al suo dovere di promuovere questa azione.

di barche a vela con piccoli gruppi di immigrati che vengono dai più diversi Paesi) dimostrano come tutto il bacino del Mediterraneo può essere il potenziale luogo di sviluppo di flussi enormi di immigrazione che, se non prevenuta e se non controllata nei Paesi di origine e di destinazione con una seria politica di sviluppo, vedrà l'Europa e l'Italia obbligate solamente ad una politica di reazione, di difesa, di sicurezza, di protezione, che non è la ricetta giusta, a mio avviso, per parlare di Mediterraneo. Abbiamo avuto quindi delle risposte dall'Unione europea, ma credo che sia il momento - e ne ho parlato con alcuni degli interlocutori, di cui vi dirò tra un istante, durante una visita in Giordania e in Siria, l'altro ieri - di dare vita ad un vero e proprio piano Marshall europeo per venire incontro a Paesi le cui economie hanno subito danni gravissimi per effetto delle ultime rivoluzioni pacifiche. Credo che non sia inconciliabile - anzi, al contrario - parlare di democrazia e di diritti da un lato, e di sviluppo economico dall'altro: le due grandi missioni devono andare insieme. Ecco perché, parlando di un piano Marshall, ritengo che si debba parlare dello sviluppo, della prosperità, del rilancio dell'economia; penso altresì che ciò debba farlo l'Europa insieme al suo alleato storico più importante, gli Stati Uniti d'America, per una volta guidando il processo e non essendo guidata. Sarebbe una grande occasione per l'Europa guidare un processo di transizione che ognuno dei Paesi interessati gestirà con le sue forze, senza interferenze, senza paternalismi, lasciando all'Europa di promuovere lo sviluppo, la crescita economica, il rilancio dell'economia. Questo sì è un obbligo e un compito che sentiamo di volere assumere. Onorevoli senatori, ho voluto subito dare alla Tunisia, nel momento dell'emergenza,

immediatamente un aiuto d'emergenza alla Tunisia: 5 milioni di euro per fare fronte ad alcune emergenze drammatiche di un Paese che è stato attraversato dal blocco completo dell'economia per alcuni giorni. Si tratta soltanto di un simbolo, di una prima azione immediata di sostegno economico, a cui ho ritenuto di aggiungere un'altra proposta di breve termine, ma anche di medio termine: l'apertura di due linee di credito finanziario alla Tunisia, per un ammontare totale di 100 milioni di euro (una somma non insignificante), prevalentemente destinate a sostenere il settore privato delle piccole e medie imprese tunisine. finanziare e promuovere, con una linea di credito *ad hoc,* che decideremo alla prossima riunione del comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo, il rilancio il rilancio del tessuto delle piccole e medie imprese dell'economia privata tunisina. Si tratta di 100 milioni di euro che saranno anche destinati ad un sistema di prevenzione dell'inquinamento del mare e per favorire la ripresa del turismo in Tunisia, uno dei settori chiave, come sapete, dell'economia tunisina. Per essere

al loro Ministro della cooperazione e dello sviluppo, in rappresentanza del Governo (come sapete, il loro Ministro degli esteri è dimissionario, e quindi si è in attesa

per identificare azioni immediate di sostegno all'economia di quel Paese. Ho proposto al primo ministro Ghannouchi che le Regioni italiane, come sapete, già sensibili ai programmi di cooperazione decentrata, possano possano adottare decisioni immediate, magari progetti piccoli ma visibili, per usare le parole del Governo tunisino, al fine di adottare qualche provincia tunisina

dove una classe media tunisina, ben istruita ma consapevole della povertà e della disuguaglianza, ha reagito. In quelle province della Tunisia, quelle sud-occidentali, ad esempio, pensiamo allora che la collaborazione delle Regioni italiane con queste linee di credito possa essere l'apripista di un'azione internazionale che si esprimerà e si concretizzerà a marzo in una Conferenza internazionale a Cartagine, dove la comunità internazionale sarà chiamata, con il sostegno prioritario di Paesi come l'Italia, a dare un contributo alle riforme politiche, allo sviluppo economico e alla collaborazione culturale. La Conferenza di Cartagine di marzo sarà la traduzione di questo urgente esempio di azione bilaterale dell'Italia in un'azione di ampio respiro che riteniamo debba essere l'embrione di un vero e proprio piano Marshall. Abbiamo bisogno di una visione di medio e di lungo termine per affrontare questo problema. Lo dico, perché il tema è fortemente sentito in altri Paesi che meno della Tunisia sono stati attraversati dalle rivoluzioni pacifiche di queste settimane. Ho incontrato il presidente della Siria Assad e il re di Giordania: entrambi mi hanno parlato in modo sincero di una frattura tra i vertici politici e le popolazioni. Questo, a loro avviso, è stato

la guida politica dei Governi con le popolazioni è stata, a mio avviso apprezzabilmente, la linea guida annunciata dal presidente Assad e dal re di Giordania, che mi hanno parlato di iniziative già decise, quali il riconoscimento dei partiti politici e l'adozione di leggi nazionali sulla libertà di riunione e di associazione anche in luoghi pubblici: quello che, in altri termini, serve per consentire l'espressione dei diritti di libertà, a cominciare dall'autorizzazione ad utilizzare tutti i mezzi di tecnologia delle comunicazioni più moderni, YouTube, Facebook e, ovviamente, l'accesso illimitato a Internet. Queste sono idee e sviluppi che si dovrebbero tradurre in tempi estremamente rapidi in riforme,

del Mediterraneo e del Medio Oriente. Con i due leader abbiamo poi parlato del patto di stabilità, sicurezza e prosperità per il Mediterraneo. Entrambi hanno manifestato grande interesse anche per una proposta che ho avanzato, quella che l'Europa promuova una progetto euro- Mediterraneo per la circolazione dei giovani, degli studenti, dei giovani professionisti secondo il modello che l'Europa ha conosciuto con Erasmus per molto tempo e che è, invece, molto ostacolato dalla regolamentazione dei visti che è in vigore nell'area Schengen per gli spostamenti verso Paesi della riva Sud del Mediterraneo. Sono iniziative su cui dobbiamo lavorare,

Il Primo Ministro e il Re di Giordania hanno sollecitato, in modo particolare, l'azione dell'Italia e dell'Europa, ho già informato ieri pomeriggio il senatore Mitchell (inviato del presidente Obama per il Medio Oriente) e che oggi affronterò con il Ministro degli esteri russo,

per non dimenticare che la pace tra palestinesi e israeliani rimane una priorità nell'agenda internazionale. Non bisogna dunque dimenticarlo, perché queste situazioni di crisi rischiano di distogliere l'attenzione

poi parlato dell'Egitto. I miei contatti con il vice presidente Souleiman e con il segretario generale della Lega araba Amr Moussa si sono intensificati negli scorsi giorni in preparazione di una mia visita al Cairo che stiamo organizzando a breve e a breve e che mi consentirà anche un incontro diretto con il ministro della difesa Tantaui per conoscere le loro valutazioni sui tempi e sulle modalità della riforma costituzionale. Il Segretario generale della Lega araba mi ha riferito che il comitato per le riforme costituzionali che, come sapete, è presieduto da un giurista di grande reputazione (l'ex Vice Presidente del Consiglio di Stato egiziano) ha ricevuto il mandato di completare gli emendamenti costituzionali in 13 giorni e di preparare il *referendum* popolare sulle modifiche costituzionali nei prossimi tre mesi. Tempi davvero rapidissimi. Bisognerà seguire con grande attenzione questo passaggio e questa fase di questa fase di transizione, che dovrà includere a mio avviso, come il ministro Tantaui ha già detto, il rispetto da parte dell'Egitto dei trattati internazionali e regionali di cui è firmatario, incluso, ovviamente, il trattato di pace con lo Stato di Israele. Sapete che questa era una delle domande che non avevano trovato chiara risposta; ora hanno trovato chiara risposta, e noi ne prendiamo atto con soddisfazione. Stiamo seguendo il dialogo con le forze dell'opposizione. Cominciano ad emergere delle candidature per le future elezioni in Egitto, che si dovranno tenere, credo, alla luce della *road* *map* presentata, tra il mese di agosto e il mese di settembre. Anche con le autorità dell'Egitto ho parlato della necessità di un piano Marshall internazionale. Pensate che in queste settimane di rivoluzione pacifica l'Egitto ha subito nella sua economia un danno superiore ai sei miliardi di dollari, una cifra enorme che ha messo davvero in ginocchio la sua economia. Credo che un'azione internazionale urgente - lo abbiamo chiamato piano Marshall per dare l'idea della mobilitazione internazionale in aiuto alla transizione democratica - debba essere immediatamente messa in cantiere. Vi posso dire che nel mio ultimo colloquio di due giorni fa con la signora Clinton ho raccolto un grande interesse e un grande favore degli Stati Uniti d'America verso l'idea di un piano economico mediterraneo di sostegno alle economie di questi Paesi. Sono molto preoccupato per la situazione economica egiziana: c'è una nuova ondata di scioperi che sta paralizzando molte aziende egiziane; è stata rinviata la riapertura delle banche e della borsa; ogni giorno che passa le località turistiche dell'Egitto restano vuote. A fronte di decine di migliaia di posti per turisti nelle località egiziane egiziane di mare più famose, solo poche decine di turisti sono andati in questi giorni a passarvi un periodo di vacanza. Vi è un altro problema, che è anche italiano, e di cui devo condividere con il Senato qualche brevissima preoccupazione. Abbiamo ricevuto un appello forte dalle autorità egiziane, egiziane, ma soprattutto da quella rete di aziende, anche italiane, del turismo, che hanno parlato di 12.000 lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro, perché le località di Hurgada e di Sharm El Sheikh sono vuote da qualche settimana. Stiamo riflettendo seriamente su una iniziativa da prendere per chiedere garanzie adeguate come, ad esempio, un'assicurazione dei *tour* *operator* e, in cambio, rimuovere quelle indicazioni di allerta, quelle indicazioni di allerta, di sconsiglio che hanno indotto il Ministero degli affari esteri a scrivere finora che non è consigliabile recarsi in Egitto. Credo che il popolo egiziano meriti un gesto d'amicizia.

Ma se vi fosse un margine, credo che questo gesto di amicizia da parte dell'Italia sarebbe straordinariamente apprezzato, ma anche utile per aiutare la ripresa di un'economia egiziana che rischia davvero, con il turismo, di crollare.

Avremo l'occasione di riunire un *forum* mediterraneo più allargato: avremo anche l'Egitto, la Turchia e la Grecia, oltre al «5 più 5». Faremo il punto sulle iniziative non di emergenza ma di visione sul Mediterraneo, affinché questo patto mediterraneo possa veramente essere lanciato. Un'ultima parola desidero dedicarla all'Iran, che è attraversato in queste ore da legittime aspirazioni di libertà di masse di popolo iraniano che chiedono di poter manifestare, che chiedono diritti, che chiedono, evidentemente, la garanzia di poter esprimere il loro pensiero. È evidente che noi sosteniamo le legittime aspirazioni di questo popolo iraniano che scende in piazza in modo pacifico. Abbiamo visto purtroppo la morte di una persona, ma la grandissima massa che si riversa nelle piazze e nelle strade sta manifestando in modo pacifico, chiedendo diritti e libertà, aspirazioni che credo dobbiamo assecondare, facendo presente ad un Paese che è uno Stato sovrano, l'Iran, che noi evidentemente ci attendiamo da parte del regime che il diritto di manifestare, che il diritto di esprimere il proprio pensiero sia garantito e che soprattutto mai vi siano repressioni repressioni della polizia nei confronti dei manifestanti. Ecco allora il messaggio che ho trasmesso ad una delegazione parlamentare che ho incontrato questa mattina: un messaggio chiaro, che evidentemente mi è sembrato doveroso trasmettere direttamente. È una delegazione invitata dal Parlamento italiano, che ho ritenuto di incontrare per aggiungere al messaggio del Parlamento il messaggio del Governo. Parlamento e Governo insieme abbiano oggi espresso a questa delegazione iraniana l'auspicio che i manifestanti siano rispettati, che i leader dell'opposizione siano garantiti, che quelle orribili minacce di condannare a morte i capi dell'opposizione, eminenti personalità politiche dell'Iran, non si traducano, non dico in atto, ma neanche in azioni concrete dirette a minacciare la vita dei leader dell'opposizione iraniana. L'abbiamo detto con rispetto, ma l'abbiamo detto con chiarezza. Credo che questo fosse il dovere dell'Italia, e continuerà ad esserlo.

Presidente, signor Ministro, abbiamo constatato che gli accordi bilaterali forse sono l'unico strumento che dà qualche risultato concreto. Infatti l'ultimo Accordo Italia-Libia a noi sembra che abbia impedito tante partenze di clandestini, o meglio abbia fermato tanti clandestini, al punto che la problematica dell'immigrazione clandestina sembrava ormai cosa quasi del passato. Questa dovrebbe essere la formula da riprendere, e a noi è sembrato che il ministro Maroni, nelle sue affermazioni sulla cooperazione di polizia, abbia voluto ripercorrere sostanzialmente questo solco. L'alternativa l'abbiamo sotto gli occhi: ci siamo noi, la Spagna, la Grecia e Malta, che subiremmo sostanzialmente un'autentica invasione. I problemi che si pongono ora, secondo noi, forse sono ancora più delicati, perché oggi dobbiamo pensare alle persone che arrivano sotto un ventaglio di ipotesi. Arriveranno clandestini, arriveranno persone che meriteranno lo *status* di rifugiato politico. Siamo preoccupati però per quei 10.000 criminali comuni evasi dalle carceri tunisine sotto la rivoluzione, che inevitabilmente arriveranno mescolati tra tanti altri. Questa è una sollecitazione ad essere estremamente accorti.

già da oggi desta grandi dubbi e particolare preoccupazione. Nel 2006 abbiamo stretto forti rapporti commerciali con la Libia.

Non parliamo di armi di poco conto: si produrranno aerei ed elicotteri di una certa rilevanza. L'accordo è tra una società libica e la nostra Finmeccanica,

signor Ministro, per limiti di tempo affronterò solamente due questioni.

ma questo non è un buon motivo per gridare all'emergenza né per paventare 80.000 sbarchi; inoltre, ho trovato del tutto fuori luogo, nel merito, nei toni e nel contenuto, la polemica con l'Europa, un *evergreen.*

Ahimè, la stabilità l'avevano anche prima, esattamente quella che hanno tentato di rovesciare. Quel che ha mosso milioni di persone è l'aspirazione alla libertà. E se non riconosciamo che questo è il valore universale che muove le genti (come muove noi, muove anche loro), che non c'è un'eccezione araba alla democrazia e alla libertà,

Però io credo che la dimensione della crisi che abbiamo di fronte necessiti per lo meno una politica europea. Quindi, le azioni bilaterali non sono sostitutive di una politica europea, che è, quella sì, effettivamente carente. Sicché, libertà, democrazia, Stato di diritto: o aiutiamo anche in questi ambiti e sosteniamo con forza certi principi, oppure credo che ogni altra scorciatoia puramente economicista non

Eppure questa piccola terra ha il cuore grande, un cuore che purtroppo fatica, perché non ha più la linfa vitale della sua economia, della sua vera economia, economia, che, se continua così, verrà distrutta. Abbiamo un grande problema sociale. Mancano le scuole e i presidi ospedalieri. Per partorire bisogna prendere l'aereo e andare a Palermo. Il costo del gasolio sta mettendo sul lastrico i nostri pescatori. Ma io sono fiduciosa sull'operato di questo Governo e, soprattutto, del ministro Maroni, sostenuta dal mio Gruppo parlamentare e dai miei concittadini. Purtroppo la situazione può degenerare. Sono ancora troppi gli immigrati sull'isola. Io sono una mamma, e sono molto preoccupata. Non capisco perché mia figlia, ancora piccola, debba restare chiusa in casa, mentre gli immigrati tunisini girano a centinaia per Lampedusa.

Soprattutto le più giovani hanno paura di uscire, nel pomeriggio o la sera, per la presenza così numerosa degli extracomunitari.

non si sa mai cosa potrebbe accadere. Lampedusa sta per esplodere. Ci sono quasi 2.000 immigrati che entrano ed escono liberamente dal centro di accoglienza. Ecco perché rivolgo l'ennesimo appello a tutti e, soprattutto in questa occasione, all'Unione europea, che si deve fare carico di questo fenomeno. Per dare accoglienza agli extracomunitari ci vogliono risorse,

Sta arrivando l'estate, e non ci possiamo permettere disdette di turisti, perché la nostra economia si basa sul turismo e sulla pesca. Ma i lampedusani stiano tranquilli, perché io lavorerò e lotterò per combattere questo fenomeno.

un concetto che lei ha espresso e che mi sembra meritevole di un minimo di approfondimento, anche perché quanto detto dalla collega Bonino

perché una volta acquisito il diritto a non essere poveri, una volta compreso che la povertà non è un destino ma una congiuntura

appena un mese e mezzo dalle prime rivolte in Tunisia, 30 giorni dall'abdicazione del Presidente Ben Ali e una settimana dalla deposizione di Mubarak, nel frattempo sono scoppiate rivolte in Algeria, Libano, Yemen, Nigeria, Marocco, Sudan, Turchia Libia (l'abbiamo ascoltato ieri), Albania e più di 5.000 immigrati affollano le coste siciliane. Lei, Ministro, giustamente è presente in Senato a riferire per la seconda volta sugli intendimenti del Governo in questa materia. Lo dico in modo ironico, perché

Visto che fino ad oggi non l'abbiamo mai fatto, almeno un intendimento c'è. Vediamo poi quando dalle parole si passerà ai fatti. Lei parla di finanziare le piccole e medie imprese della Tunisia,

Vorrei però sapere che cosa ha fatto il Governo per le piccole e medie imprese italiane, in Italia; che cosa ha fatto il Governo per il turismo in Italia.

Mi ricorda tanto quel personaggio che dove andava diceva «A Fra' che te serve?». Quello non ci interessa. Ci interessano le cose vere, non gli spot pubblicitari,

Questo, credo che sia invece il problema più serio: non ascoltano la nostra politica estera, perché non c'è una politica estera. C'è più una politica personale per gli affari del nostro - anzi, del vostro

cosa ben diversa dalle iniziative immediate per fronteggiare l'emergenza degli sbarchi di clandestini o dei capovolgimenti politici nella sponda Sud del Mediterraneo.

L'unica iniziativa degna di una progettualità appare quella del cosiddetto Piano Marshall per il Mediterraneo, nel quale intende coinvolgere, a quanto ho capito, anche l'Europa e gli Stati Uniti. Tuttavia mi permetta una riflessione: il Piano Marshall originale, di cui l'Italia beneficiò 60 anni fa, aveva un portato sì economico ma ancora di più politico. Sappiamo benissimo tutti che l'erogazione di finanziamenti da parte degli Stati Uniti era finalizzata, in una logica di Guerra fredda, a mantenere al governo dell'Italia un partito di centro ed evitare la vittoria della sinistra. qual è il progetto politico che sta dietro questo nuovo Piano economico che lei propone per il Mediterraneo? Ritorniamo di nuovo alle frasi, alle parole: io vado, io faccio. Poi, però, quando lei va lì, nessuno se lo fila! Questo è quello che abbiamo visto fino ad oggi. Le sue parole hanno ingenerato in me un'ulteriore confusione. Non ho capito, infatti, se l'erogazione di aiuti finanziari sarebbe subordinata all'instaurarsi di governi democratici, al riconoscimento dei diritti civili e politici alla tutela della libertà di espressione e della parità tra uomini e donne, come chiede l'Europa e come pretendiamo dal Governo iraniano. Oppure se, al contrario, saremmo disposti ad erogare tranquillamente i contributi anche a regimi illiberali che chiudono gli immigrati in campi di concentramento nel deserto, che negano un pluralismo politico e che predicano un islamismo militante (cosa che abbiamo fatto con la Libia). Ad accrescere ancora di più Ad accrescere la mia confusione sono stati anche gli elogi fatti dal Presidente Berlusconi a Mubarak proprio poche ore prima che fosse deposto da un popolo che anelava libertà. A me pare che il progetto politico del Governo non esista, l'ho detto all'inizio e lo confermo, ne parlano gli altri; ne ha parlato anche l'Europa. Un commissario vi ha detto: «Ma che state dicendo che l'Europa non vi sta dando una mano, se siete voi che non l'avete voluta, mentre noi ve l'abbiamo data?». Leggendo queste cose, la confusione aumenta ancora di più. Il progetto politico del Governo non esiste, e fino ad adesso l'unica seria preoccupazione che ci guida nella nostra politica estera è quella di evitare lo sbarco di clandestini erigendo muri sotto la Sicilia, o di piazzare i nostri prodotti all'estero.

sia un caso se la Tunisia ha avanzato la richiesta di 5 miliardi per riprendersi dalla crisi e bloccare la partenza dei barconi degli immigrati, in quanto 5 miliardi sono proprio quelli dati dal nostro Paese a Gheddafi. Non so se ricorda anche questo, un'altra tangente per non avere degli sbarchi in Calabria, Puglia, o Sicilia. Continuiamo noi a pagarla, non con la politica internazionale, non con le idee, ma con il denaro. Adottando una politica bilaterale basata su meri accordi economici, il nostro Paese si sta rendendo, oltre che poco affidabile agli occhi dell'Unione europea, anche ricattabile dai Paesi del Mediterraneo, perché continuiamo a dare questa

ma dal futuro del Mediterraneo. Stabiliamo innanzitutto che il nostro ruolo non può essere altalenante: non possiamo essere per la libertà e l'uguaglianza ad intermittenza così come non possiamo essere europeisti ad intermittenza, pena di essere estromessi dall'Europa che decide. L'incidente

come ha annunciato il Ministro e riprendendo le fila del processo di Barcellona; ripianare i tagli fatti alla cooperazione allo sviluppo; incentivare una cooperazione europea con i Paesi d'origine delle migrazioni, aprendo veri e propri centri europei per l'impiego nei Paesi del Mediterraneo al fine di qualificare, sul fronte occupazionale e della formazione professionale, i migranti; rivedere l'impianto della legge Bossi-Fini adeguandola alle norme comunitarie; sostenere i movimenti popolari democratici dei Paesi interessati dalle tensioni; e infine e soprattutto abbandonare la politica unilaterale di sostegno incondizionato a Gheddafi, dopo le indiscrezioni dell'AISI per cui sarebbe stata proprio la Libia ad aprire ai clandestini le frontiere con la Tunisia per evitare un effetto domino delle contestazioni su Tripoli, dopo i 38 feriti negli scontri di questa notte a Bengasi, Se l'Italia non rivede la sua politica estera ho paura che il pericolo prossimo non sia rappresentato dagli ottantamila immigrati che affolleranno le nostre coste, ma dal fatto che

con questi Paesi, bisogna ragionare in modo collegiale e non personale: lei sta ragionando, purtroppo, come fa il suo Presidente del Consiglio, in modo personale, e dell'Italia non gliene frega niente.

Credo che la situazione nel Nord-Africa sia addirittura esplosiva. Arriveranno di qui a poco i fuoriusciti dall'Egitto - lei ne ha già annunciati alcuni - dove alcuni - dove la dura rivolta della piazza ha stravolto completamente gli equilibri politici in atto da ben 30 anni, con la cacciata di Mubarak e il passaggio di poteri alle Forze armate. Quindi, arriveranno dall'Algeria, anch'essa attraversata da un fortissimo malcontento,

dove alcuni gruppi di opposizione hanno proclamato per domani la cosiddetta giornata della collera, destando forti preoccupazioni in Gheddafi; senza contare i Paesi come il Marocco, finora l'unico dell'area risparmiato dall'ondata di proteste, ma che, come la Tunisia, sta vivendo un momento difficile sotto il profilo economico, dove sono state annunciate manifestazioni per la prossima settimana. Ci sono infine il Senegal, la Nigeria. In questi Paesi, il potenziale migratorio - non lo dimentichiamo - è molto forte perché è elevata la presenza di giovani pronti a partire se le condizioni di vita nel loro Paese non miglioreranno. Tutto ciò allora produrrà ulteriori e gravi problemi di accoglienza, soprattutto, oltre ad avere pesanti conseguenze sull'economia. Lei parla di piano Marshall, che io condivido,

rivolgendosi al mercato cinese piuttosto che a quello europeo e americano. Questo non potrà che far aumentare a dismisura i prezzi nel nostro Paese, perché non può sfuggire l'utilità di materie prime come il rame e il petrolio, e di cereali, come la soia, i cui prezzi, che già oggi hanno raggiunto nuovi record sono addirittura destinati a salire. Forse non abbiamo bene vigilato sui patti bilaterali, forse non abbiamo vigilato a sufficienza su quell'Unione dei Paesi del Mediterraneo, forse non ci siamo fatti sentire a sufficienza. Certo è che l'economia globale deve prepararsi a fare i conti, nel bene e nel male, con l'onda rivoluzionaria che sta attraversando il Nord Africa e che potrebbe ora diffondersi in tutto il mondo arabo. Al problema migratorio si sommeranno forti rischi economici, rischi che in un momento di crisi economico-finanziaria come quello attuale non possiamo permetterci di correre. Quanto all'invasione tunisina, voglio dare all'atto al ministro Maroni di essersi mosso nella maniera corretta al verificarsi dell'emergenza, battendo i pugni sul tavolo dell'Europa, che è ancora una volta la grande assente. Il Ministro si è attivato mediante l'invio di uomini e mezzi, riaprendo anche il centro di prima accoglienza di Lampedusa e proponendo l'invio di agenti in ausilio. Ma se questo è vero, non posso non rilevare quanta poca credibilità ed autorevolezza abbia oggi il nostro Paese, sia agli occhi della Comunità europea, sia rispetto alla Tunisia, che rifiuta addirittura l'aiuto di uomini e mezzi. Lei parlava prima di una sorta di *feeling* con il Primo ministro tunisino.

Mi chiedo allora che fine ha fatto il patto bilaterale stilato nel 1997, che lei oggi dice giustamente di voler rinverdire, che prevedeva, tra l'altro, un dialogo permanente su queste e su altre questioni, relativamente ad una politica comune sul fronte economico, ma anche socio-culturale. Oggi lei annuncia un tavolo di confronto tra imprenditoria ed esponenti del Governo tunisino. Ben fatto. Questo tavolo è in programma per domani, ma non c'è dubbio che l'imponente esodo che ora definiamo emergenza umanitaria ci abbia colto alla sprovvista, proprio per la mancanza del dialogo previsto dal patto bilaterale. Non abbiamo vigilato, ma certamente non è stato corretto il Governo tunisino. Il confronto, che doveva essere costante e prolifico, se fosse stato mantenuto davvero vivo, avrebbe certamente aiutato a prevenire, o almeno a pianificare la gestione di questi eventi in modo adeguato. affermato dall'ex ministro dell'interno Pisanu, che sottolinea come ci siamo lasciati prendere troppo dall'ossessione della sicurezza rispetto all'immigrazione clandestina ed abbiamo perso di vista il rischio gravissimo di un vero e proprio «straripamento demografico» delle coste nordafricane? Lo stesso Pisanu rileva inoltre come il centro di accoglienza di Lampedusa sia un'ottima struttura, un centro che andava aperto subito, senza esitazioni. Chi ha pensato di tenerlo chiuso, per scoraggiare in questo modo le partenze dalla Tunisia,

Ha ragione la collega Maraventano quando afferma che l'isola di Lampedusa è stracolma di gente e non può continuare ad andare avanti così.

Inoltre, bisogna prendere atto che è stata sbagliata negli ultimi anni la politica dell'immigrazione in questo Paese: ci si è lodati per avere fermato l'immigrazione clandestina e per avere annientato gli sbarchi, sottovalutando in modo clamoroso La realtà è decisamente un'altra: l'immigrazione clandestina, stando ai dati della recentissima indagine della Caritas, è perfino aumentata nel nostro Paese, e la mole di sbarchi sotto le nostre coste è oggi sotto gli occhi di tutti. Concludendo, mi auguro che quanto proposto dal ministro Maroni circa il coinvolgimento di tutte le parti politiche su questo tema di fondamentale importanza venga concretamente realizzato e portato avanti. Per quanto ci riguarda, siamo consapevoli della gravità del problema, che non conosce e non deve conoscere colore politico, purché si tenga come obiettivo primario il fattore uomo, il fattore umano. caso, siamo disponibili ad avviare fin d'ora una collaborazione costruttiva e permanente.

Siamo chiamati ad affrontare un'emergenza che nell'opinione pubblica suscita smarrimento ed inquietudine: sentimenti naturali per qualunque popolo che avverte la precarietà o, per meglio dire, la virtualità dei confini del proprio Paese. In simili frangenti, le istituzioni dovrebbero provvedere ad acquietare i cittadini, ristabilendo la legalità con scelte ispirate a realismo e determinazione. Al contrario, parte della cosiddetta classe politica in questi giorni ha dato vita a contese verbali, a volte surreali ed inopportune. Ma i colleghi senatori del Partito Democratico credono seriamente che la gente si attenda da loro la minacciata e fantasiosa denuncia nei confronti del Ministro dell'interno per omissione di soccorso? Davvero pensano che il popolo sia turbato perché il Governo non si industria a sufficienza nell'agevolare, incoraggiare e patrocinare gli approdi delle masse clandestine?

Noi stiamo a disquisire di profughi e rifugiati politici dai Paesi del Maghreb in tumulto, ma il buon senso, che ancora abbonda tra la nostra gente, dice chiaramente il contrario. I perseguitati politici, signor Ministro e colleghi senatori, fuggono dai regimi che opprimono, non dai regimi che si dissolvono; e allora, chi ci entra in casa sotto le mentite spoglie del rifugiato? Evasi, potenziali guerrieri di Allah o volgari profittatori, che mirano a lucrare il trattamento e l'assistenza spettante ai veri rifugiati? È questo che dovrebbero spiegare i fondamentalisti dell'accoglienza indiscriminata: lo si spieghi ai lavoratori disoccupati, a cominciare dai circa 200.000 stranieri senza lavoro già presenti nel nostro Paese, categoria in crescita esponenziale. Nessuno nega l'emergenza umanitaria legata alle condizioni in cui vengono a trovarsi quanti sbarcano illegalmente. Opportunamente, il nostro Governo ha sollecitato il concorso dell'Unione europea, e opportunamente il ministro Frattini ci ha illustrato quello che intende fare oggi nello sforzo della ricezione. Sia ben chiaro tuttavia che tale contributo, anche economico, non può costituire un avallo all'immigrazione clandestina, finanziandone la stabilizzazione. Al contrario, chiediamo che questi mezzi comunitari vengano impiegati anche nel rimpatrio degli abusivi e vengano sollecitati a tale scopo, e che tutte le strategie di contrasto fin qui applicate vengano adottate con i Paesi del Maghreb, a cominciare dalle attività di prevenzione *in loco*. In conclusione, signora Presidente, non possiamo che riscontrare la fondatezza dei moniti lanciati dal nostro movimento, la Lega Nord, che ha sempre rilevato come, in difetto di un'attitudine di fermezza,

dell'immigrazione. Il senatore Bodega ha detto ora che è colpa del Partito Democratico se siamo di nuovo di fronte ad un'emergenza sbarchi. Lasciamo perdere la propaganda, senatore Bodega, la realtà è un'altra: il Governo ha finalmente capito che la questione dell'immigrazione, in particolare quella dalla costa Sud del Mediterraneo, non si risolve in solitudine ma soltanto in un contesto di forte cooperazione internazionale, innanzitutto europea. Come ha detto prima la senatrice Bonino, l'Europa non si può invocare a giorni alterni: o si crede nell'Europa e si scommette su una gestione europea con diritti e doveri, con oneri e onori, altrimenti si decide di fare da soli, magari con l'aiuto della Libia. Ci stiamo accorgendo oggi però che aver scommesso tutte le nostre carte sulla sola Libia forse non è stato - mi rivolgo in particolare ai colleghi leghisti - un affare dal punto di vista dell'interesse del Paese. Si deve allora scommettere sull'Europa e sulla cooperazione internazionale, per esempio anche quella con l'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, che più volte

Signor Ministro, noi la sollecitiamo ad un salto di qualità politica nella nostra riflessione, nella posizione dell'Italia di fronte a questa fase questa fase di cambiamento così profondo che si sta verificando nel Mediterraneo. Questa non è una crisi locale o anche solo regionale: siamo in presenza di un passaggio storico. Si usa, e spesso se ne abusa, questa espressione, ma nel caso specifico credo che questa sia la realtà. La sponda Sud del Mediterraneo, il Maghreb, i Paesi arabi nel loro insieme, stanno entrando in una fase di elevata turbolenza, di profonda trasformazione, che non può essere affrontata da un Paese come l'Italia, che è confinante con questa area strategica del mondo, a «spizzichi e bocconi», con piccole politiche, piccole decisioni del giorno per giorno, senza una dottrina, senza una visione

Parlamento) che, dal nostro punto di vista, non può non avere due pilastri fondamentali. Il primo, essenziale, è una chiara posizione dell'Italia a favore della libertà dei popoli della sponda Sud del Mediterraneo.

tuttavia, questo è un dato politico. Una grande potenza come l'Iran, così influente in quell'area, sta scommettendo sui popoli contro i regimi. Guai a noi se venissimo percepiti come quelli che stanno con i regimi contro i popoli! popoli! Questo deve essere il primo fondamentale asse della nostra politica estera. Il presidente Obama ha schierato gli Stati Uniti in maniera forte, ferma, convinta con il suo discorso storico pronunciato al Cairo nel giugno del 2009, e l'Europa deve assestarsi su questa linea. Ma l'Europa potrà farlo se l'Italia su tale questione definisce una posizione, una linea chiara. Non possiamo chiedere all'Europa di darsi una politica sul Mediterraneo, senza che l'Italia assuma un'iniziativa al riguardo. Sarebbe come se se qualcuno dei Paesi del Nord Europa chiedesse all'Italia una politica sul mare del Nord. Noi siamo nel cuore del Mediterraneo, dobbiamo essere capofila di una politica europea per il Mediterraneo e sul Mediterraneo. L'altro asse fondamentale, l'altro pilastro è certamente è certamente la questione dello sviluppo, ma anche qui ci vuole una visione, ci vuole concretezza. Stiamo attenti a promettere l'ennesimo piano Marshall. Mi consenta una battuta quasi ovvia. Il ministro Tremonti è al corrente che stiamo promettendo piani Marshall a destra e a manca? Non vorrei che poi ci trovassimo a fare i conti con i conti del nostro Stato, come è successo in altre circostanze recenti. Su queste cose non si può scherzare. È cruciale, è strategico un progetto per lo sviluppo euromediterraneo, e l'Italia deve farlo, deve essere capofila anche su questo, deve farlo con concretezza e con visione.

grato a lei e all'intero Governo per la straordinaria attenzione con la quale sta affrontando le difficili implicazioni della crisi mediterranea, soprattutto, della sponda africana del Mediterraneo. La ringraziamo perché lei ha avuto la sensibilità, in 20 giorni, di venire ben sette volte in Parlamento: due volte in Senato, due volte alla Camera e tre volte innanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato. La ringraziamo soprattutto per il pragmatismo e l'acume con cui l'intero Governo sta affrontando la crisi mediterranea, in questo supportato certamente dai sentimenti più nobili del popolo italiano e, soprattutto, di popolazioni - me lo lasci dire - come quella siciliana, che in questi giorni stanno mettendo a disposizione, con grande slancio e con la millenaria, consapevole coscienza dei loro rapporti con il Mediterraneo, strutture, uomini, volontariato ed enti locali; tutti si stanno prodigando per aiutare il Governo ad affrontare questa difficile emergenza. La ringraziamo perché lei puntualmente ci ha detto con quanta attenzione si stanno affrontando i singoli problemi, sia quelli dell'economia dei Paesi del Mediterraneo - non si può pretendere che in questo momento di confusione istituzionale si possa ragionare con degli interlocutori certi, ma si fa molto bene a cercare interlocutori affidabili

negli investimenti e nel numero grazie all'azione di questo Governo. Non per nulla nell'ultimo biennio siamo diventati il primo partner commerciale dell'Egitto e non per nulla migliaia e migliaia di piccole e medie imprese, meridionali soprattutto, sono impegnate investimenti in Tunisia e nei Paesi limitrofi. Credo che, al di là del becero e consueto disfattismo qualunquista che ha contraddistinto alcuni interventi dell'opposizione, si debba ringraziare il Governo per questa puntuale attenzione, che non è solamente all'emergenza, che è pur tuttavia improrogabile. Quando parliamo di rifugiati non possiamo parlare del dato dei rifugiati che stabilmente vengono ospitati nei nostri Paesi: 40.000 in Germania e 7.000 in Italia rappresentano il dato a regime. La senatrice Bonino ha omesso di dire che abbiamo alcune decine di migliaia di possibili rifugiati che premono sulle nostre coste e, proprio perché siamo i più prossimi, abbiamo il dovere di affrontare l'emergenza. Analogamente l'Europa ha il dovere di affrontare questa emergenza, assieme a noi naturalmente, in termini di aiuti economici, perché anche di questo vi è necessità, in termini di rafforzamento dei pattugliamenti, in termini di assistenza ai rimpatri, non prima però di aver esaminato con la nostra consueta attenzione e disponibilità umanitaria tutte quelle situazioni che effettivamente meritano il grado e l'attribuzione della qualifica di rifugiato a coloro che fuggono oggi da quei Paesi.

chiedere accordi bilaterali, cosa in cui questo Governo si è veramente espresso al meglio in questi ultimi anni. Se l'ultimo trattato è stato con la Libia,

proseguiamo in questa politica. La invitiamo a proseguire e in questo senso mi sento di poter condividere anche quanto ha detto il senatore Tonini. Proseguiamo nella *leadership* di un'iniziativa mediterranea ci compete per posizione geografica, per cultura, per storia e per interessi futuri. Ci compete guidare un'Europa distratta, molto spesso strabica nella valutazione della politica estera, perché noi ne abbiamo tutti tutti i titoli. Lo abbiamo fatto in questi ultimi due anni. Il Popolo della Libertà le è grato per l'attenzione dedicata proprio a questo flusso di interessi verso il Mediterraneo e, soprattutto, il Mezzogiorno d'Italia. Continuiamo ad essere protagonisti perché non ci si faccia illusioni. Lo abbiamo visto; da due anni a questa parte lo strabismo americano è tutto dedicato all'area del Pacifico, ad altre aree certamente importanti del pianeta, e non è escluso che anche queste turbolenze di oggi siano a causa di una disattenzione di qualcuno che, forse, negli ultimi anni, noi avevamo troppo delegato agli equilibri politici nel Nord-Africa e in tutto il Medio Oriente. Riassumiamo quindi questa *leadership* come abbiamo già fatto, continuiamo su questa strada, facciamoci promotori di quelle iniziative internazionali cui lei ha fatto cenno, dall'Unione per il Mediterraneo, che dovrebbe essere più iniziativa italiana che non francese, all'APEM, che si riunirà il 4 e il 5 marzo a Roma con la sua Assemblea internazionale, sperando che le condizioni dei Paesi aderenti possano assicurare una presenza massiccia, al «5 più 5», al CIMO, a tutte le organizzazioni che lei ha citato, ma soprattutto continuiamo nella linea politica che lei ha citato, che non è solamente di stampo economico, ma è proprio linea politica condivisione delle politiche di sviluppo, della libertà, della democrazia e quindi dell'economia in quei Paesi, così come veramente in questi anni vi siete sforzati di fare. Noi ve ne siamo grati e ve ne diamo ampiamente atto, così come crediamo

con quei Paesi. Non è pensabile che il pericolo di mutamenti istituzionali in quei Paesi possa farci allentare la tensione verso l'espansione economica e verso l'integrazione economica con quei Paesi. Checché se ne voglia dire, checché se ne possa pensare, il Mediterraneo è destinato ancora una volta nella storia del mondo a svolgere un ruolo essenziale, e noi vi siamo al centro, sia - come dicevo poco fa - geograficamente che culturalmente. Noi quindi dobbiamo assumere, così come voi state facendo, la *leadership* in quella politica.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dei commi 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 3 e del comma 3-*bis* dell'articolo 5, sui quali il parere è di semplice contrarietà. Il parere non ostativo sull'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 è reso nel presupposto che la deroga ai vincoli alle spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, operi comunque entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dal comma 5 citato. In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.1, 2.1, 5.2, 5.5 e 5.7, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

G102. come già chiesto in sede di Commissione, proponiamo al senatore Perduca una riformulazione della parte dispositiva

facendo solo due osservazioni. Il provvedimento di riordino sulle missioni è alla Camera dei deputati, quindi il Governo si impegna a concorrere, per quanto di sua competenza, in quella sede, senza adottare iniziative specifiche.

Ciò sicuramente diminuirebbe il tipo di impegno che il Governo andrebbe ad assumere, ma essendo qualcosa che è stato portato alla nostra attenzione dai diretti interessati, potrebbe dare un segnale di interesse, sia per le questioni qui sollevate sia per altre questioni che, purtroppo, non sono state incluse all'interno dei documenti presentati. Peraltro, so che anche la Lega Nord aveva altre

Presidente, l'emendamento 1.1 si rende necessario per ripristinare quanto meno l'importo erogato nel precedente semestre

Vengono distribuiti finanziamenti a destra e a manca per progetti che, alle volte, come per esempio nel caso del comma 4 dell'articolo 1, hanno a che fare con l'argomento in questione, altre volte vanno a finanziare iniziative totalmente al di fuori delle missioni internazionali (ma è questione

di una ''Casa della società civile'' a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del

dandone 300.000 al Fondo di Iniziativa adriatico-ionica che finanziamo ogni sei mesi, ma le cui attività restano abbastanza sconosciute ai più, e 1.000.000 invece per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che magari è una iniziativa meritoria.

un qualcosa che nessuno può sapere. Se infatti si va a visitare la pagina Internet del Comitato stesso, si vedrà che le attività sono aggiornate al 2009 e che si tratta per lo più di incontri o addirittura assegnazioni di premi, onorificenze, benemerenze a questo e quello. La cosa che però ritengo essere scandalosa è che il presidente del Comitato atlantico italiano è un parlamentare della Repubblica, il deputato La Loggia. Il comma 11*-bis* è stato inserito alla Camera.

Vorrei consegnare alla memoria del nostro dibattito tutto quanto, perché poi ci si meraviglia, per esempio, se la piazza tunisina o la piazza egiziana si rivoltano contro i propri tiranni, perché i soldi che si dovrebbero dedicare allo studio delle situazioni sul campo vengono usati per fare dei piaceri agli amici, i quali neanche si preoccupano di certificare il modo con cui vengono spesi. Lascio al buon senso

quando si fanno dibattiti di politica estera partecipano esclusivamente gli appartenenti alle opposizioni, all'interno delle quali le posizioni non sono uguali. Per tutte queste tutto ciò a cui si doveva prendere parte contro il Governo Berlusconi (malgrado la stampa scriva che i voti dei radicali sono ormai stati comprati dal Presidente del Consiglio), auspico che emerga il buon senso dalla parte di chi invece ritiene che alcune affermazioni stampa siano vere e - quindi - che venga fatta la richiesta di voto elettronico.

se l'intervento del collega Perduca era finalizzato a sollecitare il Partito Democratico per una aperta, evidente espressione di voto,

emendamento. Si vede che devo fare il maestrino. Essendo favorevole, e se è vero che il collega Perduca aveva bisogno di conoscere

lo sforzo complessivo sostenuto è attualmente rappresentato dalla condotta contemporanea di 28 missioni in differenti parti del mondo, per una presenza media di circa 8.537 militari impegnati quotidianamente a fronte degli 8.338 impegnati nel precedente semestre; dell'articolo, che si intende con questo emendamento sopprimere, riguarda la missione in Afghanistan, iniziata nell'agosto del 2003 in ambito ISAF, dove l'Italia, anche per coprire errori di strategia altrui, partecipa con un numero considerevole di uomini e di mezzi. Nel secondo semestre dell'anno, sarà operativo nel teatro afgano un contingente stimabile in 4.200 unità. Il precedente decreto-legge di proroga decreto-legge di proroga aveva previsto per le missioni un totale di 3.790 unità, con un'ulteriore aggiunta di 180 a partire dal 1° novembre 2010. Secondo quanto previsto dal decreto-legge in titolo, al comma 1 dell'articolo 4, è autorizzata, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 380.770.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF ed EUPOL Afghanistan. Occorre ricordare che il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata EUPOL Afghanistan alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli *standard* internazionali. Sono trascorsi nove anni dalla nostra presenza in quella regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i talebani sono sempre più forti, il traffico di droga è aumentato, i signori della guerra si sono arricchiti, dando sultanati indipendenti, la corruzione regna sovrana, le elezioni sono state inficiate da brogli elettorali di ogni genere, come è stato certificato da organismi internazionali,

alla quale era stato destinato il nostro contingente ha prodotto un fallimento, e ciò va ammesso, in ragione del fatto che tale missione ha in maniera evidente cambiato la propria natura nel corso del tempo trasformandosi in presenza militare, in violazione dell'articolo 11 della Costituzione; richiamiamo sempre al ministro della difesa La Russa. Va segnalato in tal senso che per le sole missioni ISAF ed EUPOL il nostro Governo ha stanziato, dal 2002 a oggi, oltre 3 miliardi di euro, dei quali circa il 90 per cento destinati per armamenti ed equipaggiamento, e solo il restante per interventi di carattere civile, per interventi di ricostruzione e aiuto alla popolazione. Gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnanti in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato; parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate. Va infine ricordato che il 2010 è stato l'anno più sanguinoso da quando i talebani sono stati cacciati con il contributo delle forze degli Stati Uniti e delle forze afgane, tant'è che è stato pagato un tributo in termini dì militari pari a 711 uomini e donne, di cui purtroppo 13 italiani (in

sottolineo, signor Presidente), perché non possono stare lì a combattere una guerra non loro, sotto il falso vessillo delle missioni di pace e sicuramente - come dico sempre al ministro La Russa che non riesce

voto contro questo emendamento perché ci è stato descritto un contesto ingestibile che preoccupa sempre di più dove addirittura sarebbero ormai arrivati ad essersi creati dei sultanati indipendenti nelle varie province dell'Afghanistan, e qual è la risposta dell'Italia dei Valori? Andiamo via! Direi proprio di no. Eventualmente uno resta, facendo una valutazione. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Pedica che negli ultimi otto anni non è stato guadagnato tutto quello che avremmo voluto guadagnare in termini di certezza del diritto, diritti umani, sviluppo e progresso per l'Afghanistan, ma sicuramente lo si fa mantenendo la nostra presenza militare in Afghanistan. Come ho detto durante la discussione generale, più volte abbiamo posto all'ordine del giorno dell'Assemblea la questione dell'oppio afgano. Si Si può essere contrari a prescindere, a qualsiasi tipo di guerra, e pare che per motivi elettorali all'interno del Parlamento l'Italia dei Valori insista su questa posizione. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Occorrerebbe però allo stesso tempo dare una risposta per gestire una situazione che è sicuramente sotto il controllo di pochi con delle proposte politiche. Quindi, essendo il ritiro non una risposta politica, voto contro l'emendamento dell'Italia dei Valori. Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento e chiediamo al Gruppo dell'Italia dei Valori di ritirarlo.

diversa mi pare la questione della più longeva missione di pace del mondo (risale al 1964), cioè quella delle Nazioni Unite a Cipro, che ha l'ulteriore aggravante di essere una missione dei caschi blu nel territorio dell'Unione europea.

disarmati, per controllare un cessate il fuoco iniziato nel 1964. Questa situazione, secondo me, fa il paio con i soldi dati a La Loggia, con grande interesse da parte della maggioranza e del terzo polo, che si è astenuto, quindi in sostanza è a favore di questo modo di procedere.

rappresenta - lo ripeto - la più antica missione di pace delle Nazioni Unite, che si trova con i caschi blu sul territorio dell'Unione europea (per quanto la parte settentrionale dell'isola di Cipro non sia riconosciuta da Bruxelles,

sostanza, tale ordine del giorno viene incontro alla richiesta del collega Perduca. Contemporaneamente, mi permetto di ricordare a tutti i colleghi che stiamo esaminando un decreto in seconda lettura su un tema di grande delicatezza, quello delle missioni, occorre quel necessario *fair play* che consenta all'opposizione di esprimere le sue posizioni di merito, ma anche un senso di responsabilità di fronte all'Assemblea e al Paese, in coerenza con l'importanza di questo provvedimento. Tutti siamo stati in maggioranza e all'opposizione a fasi alterne e sappiamo che ci sono dei momenti nei quali il senso di responsabilità deve fare premio.

potrebbero essere limitati. Sicuramente daremo il buon esempio, poi vedremo come ci si comporterà nel voto finale. Auspico però che anche la missione di Cipro rientri tra le trenta analisi approfondite che si faranno di qui a quando ci verrà concessa la possibilità di discutere di questo nuovo quadro

ci sono già 5 milioni di euro messi a disposizione e aggiungiamo altri 2,5 milioni di euro per fare anche delle celebrazioni nei teatri di crisi.

ringrazio il senatore Torri per avermi addirittura preceduto nella dichiarazione di voto. Quello che credo veramente non abbia né capo né coda in questo comma è che per le esigenze ivi previste anche inserite alle missioni internazionali

questi soldi avrebbero potuto essere spesi in modo migliore, magari rispondendo ad alcuni degli ordini del giorno posti in votazione poco fa o per prendere in cura

provocate da una serie di vaccini a loro imposti da parte del Ministero della difesa. La nostra Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, mi è stato detto dalla senatrice

oggi continua a far sventolare la bandiera tricolore nel mondo con orgoglio ed efficienza e che possono essere affrontati con i soldi del contribuente.

Signor Presidente, in questa sede vorrei sottolineare la coerenza del mio Gruppo. Sin dall'inizio di questa legislatura, infatti, siamo stati decisi nel chiedere al Governo di mettere a punto ed illustrare una convincente strategia d'uscita da quello che ormai possiamo tristemente definire un vero e proprio conflitto. L'Esecutivo continua a prorogare il nostro impegno in Afghanistan senza alcun criterio programmatico, senza alcuna previsione di soluzione futura, anzi aumentando addirittura il contingente. Dopo nove anni di nostra presenza in quelle regioni i risultati sono sotto gli occhi di tutti:

e stabilizzare il Paese è il covo della corruzione; la produzione di oppio è aumentata di 40 volte; il numero delle vittime civili non è mai stato tanto alto come nel 2010. Drammatiche evoluzioni a parte, chiediamo il ritiro immediato delle nostre truppe per un altro importante motivo. L'Italia dei Valori ha infatti seri dubbi sulla compatibilità del nostro impiego operativo in Afghanistan con quanto contenuto nel testo costituzionale, nello specifico con l'articolo 11 della Costituzione. Questo Governo non ripudia la guerra. Si badi bene, colleghi, che l'Italia dei Valori con questo ordine del giorno non vuole in alcun modo sostenere la necessità per il nostro Paese di uscire dalla NATO. Siamo ben consapevoli, infatti, dell'importanza storica ed attuale che discende dalla partecipazione dell'Italia alla stessa. Poniamo però, al contempo, il quesito della compatibilità delle modalità operative e pratiche di svolgimento di questa missione con il dettato costituzionale testé citato. Per questi motivi chiediamo nell'impegno al Governo che sia esso stesso a valutare, tramite iniziative diplomatiche a carattere internazionale, la compatibilità di detta missione

perché il dispositivo è assolutamente non condivisibile. Vorrei ricordare che nel famoso discorso, che ho avuto modo di citare anche alla presenza del ministro Frattini,

Dopo l'attentato alle torri gemelle, non era possibile evitare quell'intervento. Ora noi siamo in Afghanistan per garantire l'equilibrio possibile in quel Paese attraverso una strategia che non è di uscita immediata e banale. È invece una strategia che è stata definita dagli Stati Uniti d'America e dagli alleati della NATO, sempre con la piena autorizzazione delle Nazioni Unite che hanno fatto risoluzioni su risoluzioni, anno per anno, autorizzando la missione in Afghanistan, volta a procedere a una progressiva messa in sicurezza di aree crescenti del Paese dove trasferire la responsabilità della sicurezza e della difesa alle forze afgane, con il pieno consenso e con la piena collaborazione del Governo afgano, per poi iniziare gradualmente una forma di rientro che deve essere parallela alla presa di controllo da parte delle autorità afgane. Questo Questo rientro dovrebbe cominciare gradualmente già questo anno nelle aree che già sono in qualche modo messe in sicurezza e si prevede che possa concludersi nel 2014. Credo che un Paese come il nostro non possa permettersi, su una questione così seria e rilevante a livello internazionale, internazionale, delle uscite estemporanee e, men che meno, degli atti unilaterali. Siamo dentro un sistema di alleanze storico per il nostro Paese, che è uno degli elementi costituivi della nostra politica estera. Per noi non è accettabile e pensabile

delle Nazioni Unite. Il nostro voto non può che essere contrario, ma rinnovo l'invito ai colleghi dell'Italia dei Valori a ritirare l'ordine del giorno G4.100, per evitare anche una divisione politica che avrebbe caratteristiche non ordinarie, data la rilevanza della materia.

nessuno mette in discussione né le nostre alleanze né la nostra collocazione internazionale.

Signor Presidente, mi è sembrato doveroso, al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che a seguito di missioni abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, comprendere l'esposizione all'uranio impoverito e soprattutto alle nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. La convinzione dell'importanza di questa precisazione mi viene dalle numerose sollecitazioni pervenutami dai familiari dei ragazzi deceduti e soprattutto da una sentenza del TAR di Napoli e dalla relazione presentata in Commissione dalla dottoressa Gatti, ricercatrice dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che da oltre dieci anni sta studiando gli effetti delle polveri inorganiche

Una spiegazione del tutto possibile è legata all'esplosione di bombe ad alta tecnologia e segnatamente quelle all'uranio impoverito, al tungsteno ed altre di nuova generazione che si caratterizzano per l'elevata temperatura generata (oltre 3.000 gradi). Il calore fonde il bersaglio e in parte lo vaporizza, generando così degli aerosol di polveri sottili ed ultrasottili. L'inalazione o l'ingestione di cibi contaminati da queste polveri immette nell'organismo processi flogistici che generano tumori, perché è ovvio che la circolazione porta queste polveri in tutto il corpo, compresi linfonodi, gonadi e cervello. Molti reduci hanno sviluppato tumori ai testicoli e le loro compagne sono state colpite dalla cosiddetta "malattia del seme urente". Nel giugno scorso la dottoressa Gatti è stata invitata dalle autorità statunitensi competenti ad un *workshop* della NATO per presentare un seminario dal titolo «Nanoparticelle: una nuova forma di terrorismo?». Vogliamo una volta tanto pensare seriamente a tutti quei ragazzi che hanno perso la vita e alle loro famiglie che ancora li piangono e non sono state minimamente indennizzate?

aveva fatto cenno, nell'ambito della relazione, al fatto che sia stata introdotta da parte dell'altro ramo del Parlamento, attraverso un emendamento che è recepito nel testo, una migliore formulazione dell'articolo del codice dell'ordinamento militare che fa riferimento al riconoscimento delle cause di servizio, prevedendo una forma più ampia, tale da consentire più facilmente il riconoscimento di questa causa di servizio e quindi dei relativi indennizzi anche per le situazioni cui esplicitamente fa riferimento la proposta di emendamento. Non posso escludere che questa indicazione esplicita possa in qualche modo ulteriormente favorire l'obiettivo perseguito anche se per la verità ho qualche dubbio, perché la formulazione, così com'è stata predisposta in sede di emendamento approvato dalla Camera, mi sembra già sufficientemente comprensiva, perché in realtà qui si vuole in qualche modo sottolineare quello che peraltro dovrebbe già essere compreso. In ogni caso, atteso il fatto che anche un eventuale inserimento di questa dizione comporterebbe - com'è noto - il ritardo nell'entrata in vigore della legge di conversione, ritengo di poter formulare un invito al ritiro alla senatrice proponente dell'emendamento 5.8, proprio nel senso di condividere l'auspicio e l'obiettivo, ma non di far sì che alla fine, per qualche precisazione o maggiore inserimento di tipo lessicale, si finisca per non ottenere proprio il risultato voluto. Eventualmente penso possa essere esaminata la possibilità di inserire questo tipo di aggiunta in qualche altro veicolo legislativo che non metta in difficoltà l'approvazione definitiva del provvedimento e quindi anche l'entrata in vigore di quella norma che comunque è già

Secondo i nostri studi, infatti, si potrebbe arrivare a risparmiare fino a 30 milioni di euro eliminando alcuni privilegi che restano in capo a ex rappresentanti dell'Esercito o di altre istituzioni, ivi compresi i rappresentanti del Governo, relativamente alle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione. Mantengo quindi gli altri emendamenti, che avrebbero voluto ampliare

proposte e approvate dalla Camera dei deputati all'articolo 603 del codice dell'ordinamento militare hanno ampliato la platea delle persone che, per causa di servizio, dovrebbero avere degli indennizzi adeguati. Questo riguarda il personale italiano.

che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità, allargando la platea

dell'intervento della Camera e anche della nostra eventuale approvazione. aggiungere la mia firma all'emendamento 5.8, che diventerà un ordine del giorno, e ricordo al Governo che tra le varie patologie tumorali sulle quali, opportunamente, si cerca di intervenire,

dare una migliore definizione dei danni biologici gravissimi, che arrivano fino al decesso, che riguardano personale militare e civile, però è compito anche del Parlamento prevedere una idonea copertura, perché

e si impegna a valutarne l'inserimento in atti discendenti amministrativi, a seguito dell'approvazione di questo provvedimento, al fine di valutare correttamente sia l'esposizione all'uranio impoverito che, per quanto è stato ricordato, al radon.

Presidente, l'intervento del collega Tonini ha ulteriormente, come altre volte, nobilitato la discussione

su un ennesimo emendamento identico, che riguardava l'esimente per i nostri militari, abbiamo chiesto che venisse indicata con chiarezza la catena di comando e venisse incardinata la questione nel codice penale militare. Il motivo è legato al fatto che la grande professionalità dei nostri militari è dovuta anche alle responsabilità che esercitano i comandi. Pertanto, non è possibile affidare un'esimente semplicemente alle regole di ingaggio.

ricordato a sua volta nell'intervento che ha testé concluso, due specifiche norme di questa natura sono state introdotte proprio dall'Aula del Senato, in occasione della conversione di un precedente decreto

una definizione delle normative penali militari è stata condivisa trasversalmente dal Parlamento, e quindi da entrambi i rami

che, per varie ragioni, non sono arrivati a conclusione nei tempi di esaurimento delle rispettive legislature. Certo, l'esigenza più sentita è ovviamente quella della definizione delle norme penali militari che concernono gli attuali impieghi nell'ambito delle missioni internazionali, che sono di maggiore delicatezza perché, per semplificare, non possono essere riferiti con

innovative e di grande rilievo per l'epoca nella quale furono emanate, ma che certamente non si attagliano perfettamente alla situazione attuale. il Governo hanno comunque già operato in questo senso. Rispetto agli impegni precedenti, è stato presentato un disegno di legge da parte del Governo sulla predisposizione di un nuovo codice penale militare riferito alle missioni internazionali, il quale al suo interno vede, tra le principali questioni, quella a cui fa riferimento

trovano sede nello stesso provvedimento a cui facevo testé riferimento.

a me pare abbastanza chiara) è di arrivare alla vigilia del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale portando a termine il processo legislativo già incardinato

implementassimo (uso un pessimo anglicismo) o adeguassimo il nostro codice penale alle norme contenute in quello Statuto, molti dei problemi che ci portiamo avanti relativamente alle responsabilità penali dei militari nostri e altrui

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2537, impegna il Governo ad adoperarsi, nei limiti di competenza, affinché l'interpretazione del comma 3*‑bis,* lettera comma 1, ivi sostituito, possa ricomprendere l'esposizione all'uranio impoverito e alle nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, nonché l'esposizione al radon».

Quindi, mettere al primo punto la cooperazione e successivamente il rifinanziamento delle missioni non corrisponde al vero. Tuttavia, ci rendiamo conto di molte delle cose che qui sono state dette. Con lo spirito che poco fa fa animava il senatore Di Giovan Paolo, mantenendo la sua posizione rispetto agli impegni che abbiamo fin qui assunto, anche rispetto a questa

impegni il Governo a definire, per l'atto di proroga futuro del rifinanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione internazionale, un titolo nell'ordine dei termini effettivamente corrispondente alla prevalenza della spesa.

- e l'elemento che riguarda il titolo lo disvela - sia finalmente oggetto di attenzione maggiore da parte della nostra Aula: questo valga per il futuro. Mi ha molto colpito in questo pomeriggio

ovviamente è una questione su cui deve esprimersi il Governo, e comunque se ne riparlerà alla prossima occasione. A me sembra un emendamento, così come l'ordine del giorno, un po' mercatistico: l'importanza di questo provvedimento non è quanto si spende per fare una cosa o quanto non si spende per farne un'altra. L'importanza di quello che si fa non è solamente legata a quanto si spende: ci sono cose molto importanti per cui si spende di meno e - ahimè - cose che possono anche apparire meno importanti per cui si spende di più.

della mia dichiarazione

le opportune azioni legislative affinché il Parlamento non sia continuamente impegnato ad approvare questi rifinanziamenti. Per queste attività internazionali sarebbe possibile ed auspicabile prevedere un finanziamento annuale, visto il continuo impegno di tempi e risorse parlamentari che si sottraggono ad altri provvedimenti non è di alcuna utilità, sia al Paese che al funzionamento delle istituzioni.

Presidente, Sottosegretario, colleghi, il provvedimento all'esame oggi concerne la proroga fino al 30 giugno di una moltitudine di interventi militari ed umanitari

il sostegno al Governo anche in questa circostanza e si stringe, una volta di più, intorno ai militari che rappresentano per il nostro Paese un grande orgoglio in un contesto tanto difficile, esponendosi a gravi pericoli che tutti conosciamo. A loro va tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro convinto apprezzamento, per il coraggio e l'abnegazione dimostrata e la professionalità nel loro operato. Alle famiglie dei caduti rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ed a quelli dei feriti auguriamo un pronto e pieno ristabilimento. Colleghi, la Lega Nord è stata senza dubbio una delle forze politiche che da sempre ha insistito sulla necessità che i nostri soldati fossero messi in una ottima condizione di difesa e di potersi proteggere al meglio. Apprezziamo che durante l'ultimo intervento del Ministro si sia parlato di stanziare i fondi per mettere in condizioni l'*intelligence* di dare una mano ai contingenti; questo è stato fatto. Prima ne ho parlato in tono polemico dicendo che secondo noi 5 milioni erano pochi rispetto ai 7 milioni e mezzo per le celebrazioni; però, è stato fatto questo e pertanto onoriamo il fatto che il Ministro abbia mantenuto l'impegno. Non possiamo esimerci dal ricordare che durante l'approvazione di questo decreto sono stati infilati all'interno dello stesso delle delle materie che poco avevano a che fare, secondo noi, con l'operato delle missioni. Ci eravamo ripromessi di non porre ordini del giorno né tanto meno emendamenti; d'altra parte devo fare le congratulazioni al al senatore Perduca che ha fatto approvare un ordine del giorno per un minimo concetto di riallineamento per quanto riguarda alcuni carabinieri. Gli fa onore e e forse anche al Governo averlo accettato. Spero che il Governo tenga fede anche ad altri

in capo ai comandanti presenti sui teatri operativi, per i cosiddetti *quick impact projects,* che servono per dare un contributo di assoluto buon senso nei rapporti con i capi delle tribù presenti nei vari territori.

di contabilità non si riesca a realizzare una legge che ci possa mettere in condizioni di sicurezza nell'approvazione dei decreti. Riteniamo inoltre che occorre avere un grande rispetto per i nostri militari dispiegati nei teatri di crisi. Come Lega, avevamo chiesto un impegno importante da parte del nostro Governo anche sulle condizioni

il presidente De Gregorio che mi sta ascoltando lo sa bene - sono stato molto critico, poiché non abbiamo messo a frutto le rendite che avremmo dovuto avere all'interno

infatti decidendo di far permanere 8.537 soldati, uomini e donne, nelle nostre missioni internazionali;

missione nei Balcani, con una decisione concordata con gli alleati; va verso la conclusione la missione «Althea» in Bosnia; abbiamo una lieve riduzione in Libano

continuiamo l'azione in Libia; prosegue l'azione di contrasto alla pirateria in Somalia; abbiamo poi stabili i presidi in Africa: Somalia, Darfur e Congo, anche se molto contenuti. Penso sia importante, tutte le volte che c'è questo tipo di passaggio parlamentare, non fare una discussione distratta o burocratica, anche se purtroppo, l'impianto del decreto in qualche modo un po' la induce. È un impianto che ancora tiene distinte la parte della cooperazione dalla parte militare, mentre si

come avremmo bisogno di decreti più fluidi dal punto di vista della normativa. Non dovrebbero esserci norme giuridiche sul trattamento del personale, proprio per poterci concentrare sul senso delle missioni che continuiamo ad approvare e che dobbiamo decidere di rivedere.

Il senatore Tonini ricordava l'importante discorso del presidente Obama e la revisione della strategia rispetto all'Afghanistan. Il presidente Obama dichiara

In molti interventi in discussione generale si è ricordato che l'Italia contribuisce molto in termini di personale e truppe per quanto riguarda le missioni internazionali: siamo appunto il quarto Paese dal punto di vista della contribuzione. Però la domanda rispetto a questo impegno così importante è: quale politica estera? Come mettiamo a frutto il fatto di essere un Paese così impegnato?

Sono stati molto limitati rispetto a ciò che sarebbe stato necessario. Come dicevo, si tratta di un atto molto importante (ricordavo il numero dei militari che inviamo perché di questo dobbiamo sentire la responsabilità),

Tutte le volte diciamo che è improprio inserire in questi provvedimenti norme giuridiche per missioni che hanno cambiato la natura di guerra o di pace

Il momento in cui ci occupiamo con più emozione, e forse anche con più attenzione (anche se non sempre), di quello che avviene nel mondo militare, almeno in Aula, è quando si registrano delle morti. Voglio ricordare che le missioni dei nostri militari all'estero sono al servizio del buon nome e dell'immagine del nostro Paese. Non so se la politica, il Parlamento, il Governo sono sempre all'altezza di questi nostri concittadini che servono la Nazione con disciplina ed onore al di fuori dei confini del nostro Stato.

il provvedimento sulle missioni internazionali è uno degli aspetti fondamentali del nostro Governo e del nostro agire. Ringrazio innanzitutto le Commissioni riunite esteri e difesa, da me presiedute insieme al presidente Dini, rilevato l'estrema importanza della proroga delle autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La concordia emersa in sede di discussione parlamentare riconferma con voce forte la valenza del contributo che l'Italia vuole assicurare nei teatri più instabili nel mondo, un contributo fondamentale, plasmato sul lodevole obiettivo di circoscrivere quelle aree suscettibili di propagare il terrorismo. Si tratta anche di un contributo volto a garantire la pace, la ricostruzione istituzionale e sociale in quei Paesi che sono riusciti, grazie all'intervento costante della comunità internazionale, a debellare il loro germe di autodistruzione. Questo è avvenuto grazie alla nostra missione, al nostro Governo, al vostro appoggio e all'appoggio di tutti i presenti.

contro le sopraffazioni dei più forti. Non è più una questione di Stati; è piuttosto una questione di uomini, donne e bambini ai quali noi dobbiamo dare democrazia e dignità. Dobbiamo, quindi, essere fieri

Dobbiamo ringraziarli perché ci hanno sempre dato grandi prove dedicandosi ai compiti loro affidati con abnegazione, costanza, determinazione e grande professionalità. Non possiamo disconoscere il loro indispensabile ruolo, in assenza del quale l'Italia non si sarebbe potuta fregiare del fatto di essere stata chiamata a far parte dei più alti consessi internazionali. Si aggiunga, inoltre, che urge coerenza tra le iniziative politiche e diplomatiche e l'azione militare, ai fini di un impiego efficiente delle risorse accordate, un altro motivo per cui il Parlamento deve ribadire il suo sostegno ai processi di pacificazione e di cooperazione allo sviluppo nonché alle missioni di lotta del terrorismo. quindi dire che la piena legittimazione giuridica è la base imprescindibile di un operato che poggia sul consenso delle popolazioni.

i Sottosegretari che sono costantemente presenti in questo scenario strategico. La buona riuscita delle missioni non può dipendere dai cambiamenti di umore della politica. È questo il campo in cui le contese partitiche devono mettersi da parte per lasciare spazio all'acume e ai ragionevoli suggerimenti dei tecnici e dei militari.

È il teatro che si pone sul piano maggiormente preoccupante. La strategia predisposta dal generale Petraeus mirante a un disimpegno militare per il 2014 richiede infatti il raggiungimento di un adeguato livello di autosufficienza delle forze di polizia e di sicurezza locali. Non dimentichiamo in questo contesto il grande valore dei nostri soldati e - lo ripeto - soprattutto dobbiamo essere deferenti per coloro che hanno perso la vita. Ultimamente altri fenomeni terroristici hanno coinvolto direttamente cittadini italiani, come il recente abbordaggio della petroliera «Savina Caylyn», nel golfo di Aden. L'alta concentrazione di attacchi da parte di pirati somali rende sempre più urgente la predisposizione di sforzi unanimi per il contrasto del fenomeno. Ovviamente non siamo soltanto in Afghanistan, ma dovremmo parlare dell'Iraq, del Libano, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Congo,

che ha prodotto un fenomeno opposto, che dovrà essere oggetto di una nostra attenta analisi, perché stiamo assistendo alla rivoluzione di Internet, di Facebook e dei *social network*. Oggi anche dai luoghi più remoti è possibile conoscere ciò che avviene nel resto del mondo. Le tecnologie mediatiche di trasmissione dei dati e la velocità con cui si propaga l'informazione digitale hanno reso effettiva la diffusione in tempo reale di messaggi di libertà. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Quindi assisteremo, nelle situazioni che si stanno evidenziando in Medio Oriente, a scenari che possiamo considerare come la caduta del Muro di Berlino del 1989. Termino

il partito che ho l'onore di rappresentare in questa dichiarazione di voto dà ovviamente il voto dà ovviamente il suo massimo apporto e voterà a favore del provvedimento per rispetto della democrazia, di coloro che operano, dei nostri militari e dei nostri caduti.

Siamo d'accordo a che esista la presenza italiana nel mondo, ma non siamo d'accordo sul modo con cui essa viene prorogata attraverso questa misura. Speriamo che l'ordine del giorno, il primo che abbiamo discusso oggi e che è stato fatto proprio dal Governo, possa segnare per la prossima volta un salto di qualità e finalmente si possa parlare di politica sulla base anche della valutazione della nostra presenza nel mondo.

si è concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Poiché l'esame dei disegni di legge nn. 2482 e connessi sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate non si è ancora concluso in Commissione, la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata esclusivamente allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

considerate di interesse generale e, al tempo stesso, utili a costituire spunti di riflessione per i colleghi in attesa della ripresa dei nostri lavori. Chi vi parla, che normalmente è solito occuparsi di giustizia, vorrebbe offrire un piccolo contributo conoscitivo ai colleghi per aiutarli a orientarsi in questa tempesta mediatica

la motivazione posta a fondamento della decisione del GIP di Milano di disporre il giudizio immediato nei confronti di Silvio Berlusconi. Voglio rassicurare i colleghi che si tratta di una illustrerò ricordando anche come il presupposto del giudizio immediato sia l'assoluta evidenza della prova.

"Quanto al delitto contestato al capo *b)*, le molteplici fonti di prove acquisite, di natura dichiarativa, documentale, intercettativa e investigativa pura, convergono nel senso della ricostruzione delittuosa prospettata dall'accusa, né, allo stato degli atti, tali esiti tali esiti probatori paiono efficacemente contrastati dai contenuti delle investigazioni difensive, che in più punti stridono in termini netti con le acquisizioni della indagine pubblica, in modo tale che la sede naturale della dialettica probatoria che già si profila è a maggiore ragione quella processuale richiesta dal pubblico ministero". In un processo di parti, quale è quello che caratterizza il nostro sistema processuale, le investigazioni difensive della difesa equivalgono alle investigazioni dell'accusa. gli elementi di prova raccolti dall'accusa stridono in termini netti con le investigazioni difensive, dov'è, onorevoli colleghi, quell'evidenza della prova che legittima il giudizio immediato? Lascio all'Assemblea

di invitare il Governo a ricevere le rappresentanze sindacali di questi lavoratori. È indecente ciò che sta avvenendo in una situazione pesantissima di crisi, a meno che

la Presidenza ancora una volta si farà carico di sollecitare questo tema che, sappiamo, ha un grande rilievo. **Sul livello

noto fenomeno del rumoreggiare, più o meno voce alta, dei senatori. Ciò però è dettato da esigenze inevitabili di comunicazione, che a volte potrebbero essere

il livello massimo di rumore previsto dalla normativa, approvata anche in questa nobile Aula, per la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Credo dunque che bisognerà trovare una soluzione diversa. Do perfettamente ragione, in particolare a lei, che è sempre solerte su questo punto, nel richiamare noi tutti, può succedere anche a me, a parlare a voce più bassa possibile quando non si ha la parola. Tuttavia, il fatto di alzare oltre ogni limite, anche di salute,

un'*escalation* che non dà beneficio, né al decoro né alla salubrità di questa Aula.